è riportata una nota della Ragioneria generale dello Stato secondo la quale vi è un peggioramento del *deficit* per il 2008.

Presidente, vorrei intrattenere per qualche momento l'Assemblea su una informazione di cui dispongo e chiedere il suo autorevole intervento presso il Ministro dell'interno per stigmatizzare, forse anche per censurare e rimuovere, il questore della città di Roma che oggi si è reso responsabile di un comportamento incivile e di vero sabotaggio di una libera manifestazione politica. Migliaia di persone sono state sequestrate sui pullman e bloccate per tre ore all'aeroporto di Fiumicino e nel tragitto da Fiumicino al centro di Roma per impedirgli di partecipare ad una manifestazione politico-istituzionale di tutti gli amministratori locali della Regione Sicilia che si svolgeva a Piazza Montecitorio, con un comportamento premeditato. Ieri, infatti, c'era stata negata la piazza e oggi, con la gestione tecnicamente perfetta delle forze dell'ordine, è stato impedito ai partecipanti di raggiungere il centro di Roma: il questore si è veramente impegnato in una operazione di sgombero politico. Siccome la questione è di una evidenza e di una gravità assolute e lei sa, signor Presidente, che ieri l'avevamo avvisata chiedendo il suo intervento, che c'è stato, chiedo formalmente che il Ministro dell'interno venga a relazionare qui in Parlamento per capire se ancora, al di là delle questioni di sicurezza che vengono utilizzate strumentalmente in casi come questo, vi sia la possibilità di manifestare liberamente in questa città

che ha permesso che interi pezzi del territorio fossero presidiati dalla malavita; un questore che non si è reso conto delle baraccopoli e della favelizzazione progressiva della città, poi impedisce una manifestazione democratica di un partito rappresentato in Parlamento. Questo questore può stare nel Venezuela di Chavez, non nell'Italia democratica: il suo è un atteggiamento intollerante.

ma ho ricevuto telefonate di alcuni manifestanti che denunciavano il comportamento della questura di Roma. Mi associo quindi a ciò che hanno detto i colleghi, affinché il Ministro dell'interno trovi il modo, nella giornata di oggi, di venire a riferire in

ma non si può mettere in discussione la democrazia e la possibilità di manifestare liberamente da parte dei cittadini italiani, perché un questore ed una questura proibiscono tutto questo. Ciò è assolutamente inammissibile.

la relazione spedita questa mattina dal Ministero dell'economia... dimostra che il Governo ha mentito al Parlamento; il Governo ha detto una menzogna al Parlamento e l'ha detta per iscritto.

Ha trasmesso un foglio di carta, spacciandolo per relazione tecnica sulla legge finanziaria, che è fondamentale per l'Italia,

come copre quanto detto dalla Ragioneria, vale a dire che la finanziaria è attualmente scoperta per oltre 200 milioni di euro. Questo è il mio intervento sull'ordine dei lavori, Presidente.

ossia che l'emendamento 3.2000 non fu sottoposto a relazione tecnica proprio perché era scoperto, e questo si evince chiaramente dalle carte trasmesse dal Ministro. Per inciso, il Ministro ieri ha detto che non c'era un problema di copertura, ma si trattava di una questione relativa all'indebitamento netto, che sarebbe un aggregato statistico: forse farebbe bene a rinfrescarsi la memoria sull'argomento. se l'emendamento è stato votato, così come risulta, scoperto, vuol dire che era assolutamente inammissibile, quindi, non si può fare i rigoristi ad intermittenza: il Presidente della Commissione non lo doveva ammettere. Aquesto punto, occorre dare una svolta seria ai nostri lavori, perché queste carte parlano chiaro: siamo davanti ad una finanziaria scoperta, nella quale si dice che in qualche modo bisogna recuperare effetti per centinaia di milioni di euro nell'ambito della discussione in Aula. La cosa in Aula è difficile da realizzare, perché gli emendamenti arrivano come un profluvio e non si possono valutare gli effetti finanziari degli emendamenti *a* *priori* per avere la certezza di compensare questo buco di 200 milioni.

sia una fonte incontrovertibile - e penso che saranno d'accordo anche i colleghi della maggioranza - ha affermato che, per effetto degli emendamenti approvati in Commissione, c'è un peggioramento del *deficit* di 94 milioni

c'è qui il Governo, il quale risponderà. No, signor Presidente, perché sull'ammissibilità degli emendamenti e soprattutto sulla loro copertura giudica la Presidenza, cioè lei, signor Presidente. Lei deve allora esprimersi sulla questione

Avete preso in giro, anche con urla e schiamazzi, i giusti richiami - e qui c'è la prova che erano giusti - del senatore Baldassarri, ma se vogliamo essere un Paese serio

Quando c'eravamo noi, voi lo pretendevate; non fate, per cortesia, che tutte le regole valgono per una stagione e poi non valgono più per l'altra. Signor Presidente, lei è supremo garante delle regole in questo ramo del Parlamento. Lei deve - questo è il mio accorato appello - farsi parte diligente perché non è soltanto suo diritto, ma soprattutto suo dovere. C'è la prova che in Commissione qualcosa non è andato per il verso giusto, la prego di intervenire.

il punto oggi evidenziato dall'allegato 7, che è stato rielaborato dopo i lavori della Commissione, era ampiamente noto durante i lavori della Commissione, tant'è che,

dei *ticket* per il 2008. L'allegato 7, da questo punto di vista, non fa che confermare, dunque, il tema di cui abbiamo discusso durante i lavori della Commissione. durante quei lavori, io ho sostenuto una certa tesi, anche prendendo per buona la posizione che a quel punto ci era nota, perché il Governo aveva depositato in Commissione lo scambio di

anche ammettendo che, in questa dialettica di posizioni diverse circa l'interpretazione dell'utilizzo per la copertura dell'emendamento *ticket* del cosiddetto Fondo Amadori per le politiche comunitarie,

un problema di inammissibilità dell'emendamento non si può proporre e non si propone perché la Ragioneria non mette minimamente in discussione questo punto - il fatto che l'utilizzo di quel fondo a fini di copertura sul lato della competenza, cioè sul lato del saldo netto da finanziare, sia perfettamente corretto.

sotto il profilo della competenza, la copertura è perfettamente corretta; la cifra che riconosce sia l'ufficio legislativo - e il Ministero in generale - con la nota tecnica depositata in Commissione è 326 milioni di euro. In Commissione, infatti, la relazione tecnica c'è; è quella depositata dal Ministero dell'economia che reca la firma del professor Sartor. In quella nota tecnica, sul versante della competenza, la copertura derivante dall'utilizzo del cosiddetto Fondo Amadori cifra 326 milioni di euro. Sotto questo profilo, dunque, non si può proporre alcun problema di legittimità e di ammissibilità dell'emendamento. L'emendamento era correttamente, secondo me, all'attenzione della Commissione, è stato ammesso e, una volta approvato, è correttamente all'esame dell'Aula, essendo stato inserito nel testo approvato dalla Commissione. Si pone, ora (e l'allegato 7, a mio avviso, utilmente evidenzia questo problema), la questione, più delicata e più controversa, sotto il profilo tecnico, di come cifrare l'effetto, sul versante della cassa, cioè sul versante dell'indebitamento netto, di quello stesso utilizzo di 326 milioni del Fondo Amadori. Da questo punto di vista, non c'è dubbio, signor Presidente, che, a mio avviso, la tesi della Ragioneria ha qualche fondamento quando sottolinea che, escluso qualsiasi escluso qualsiasi problema di ammissibilità, l'effetto di cassa di quella riduzione del Fondo è diverso, quantitativamente diverso, dall'effetto di competenza. Dunque, sul versante della cassa, secondo me, è pacifico, malgrado la posizione diversa del Ministero dell'economia, che ci sia un effetto diverso. Questo, però, signor Presidente, non vuol dire che l'emendamento era inammissibile e, non avrei dovuto ammetterlo e quindi il testo approvato dalla Commissione è inammissibile. Significa semplicemente che, come evidenzia l'allegato 7, si è aperto un problema sul versante dell'indebitamento. Sto cercando di Sto cercando di dire quello che penso, non sto facendo polemiche con nessuno. Secondo me, il problema sul versante dell'indebitamento c'è e - a mio avviso -sarebbe opportuno correggere qualcosa per tenerne conto; conto; sono convinto che sarà fatto perché deve essere fatto. Non c'è un problema di inammissibilità, ma solo il problema di correggere ciò che eventualmente si sia determinato sul versante dell'effetto di cassa.

una volta detto questo, signor Presidente, la vera questione che si pone, in quel momento, è: di quanto bisogna correggere? Di quanto l'effetto di cassa è difforme rispetto all'effetto di competenza?

che utilizzava il Fondo Amadori per un intervento sull'indebitamento della sanità, esattamente lo stesso tema: stesso problema da risolvere, stessa copertura effettuata. A dimostrazione che il tema è controverso, specie per la sua quantificazione, lo stesso Ragioniere generale dello Stato, che non è cambiato nel frattempo, ha detto che l'effetto di competenza e l'effetto di cassa coincidevano. La Commissione bilancio disse che aveva alcune perplessità su questa coincidenza, tant'è vero che un intervento successivo mise riparo, almeno in parte, a quella che allora considerai una valutazione tecnica infondata della Ragioneria. Ora, però, signor Presidente, lei mi deve scusare, ma passare in sei mesi, sullo stesso tema, pretendendo di mantenere intatta la propria credibilità tecnica, dalla tesi dell'identità di effetto competenza e cassa,

bisogna riconoscere che è questione molto controversa quella dell'effetto di utilizzo di fondi, come quello Amadori, sul lato della cassa rispetto a quello della competenza; in terzo luogo, non c'è dubbio che esiste una differenza tra tra l'effetto di competenza e l'effetto di cassa e che, in qualche misura, bisognerà porvi rimedio, non perché si pone un problema di ammissibilità, ma per mille altre ragioni. Non è vero affatto, appunto, che l'indebitamento netto sia un dato meramente statistico, ma è un dato di primario rilievo economico e finanziario; la

Su quel lato si pone un problema, mentre non esiste nessun problema di inammissibilità. Non c'è dubbio che, nel corso della lettura della finanziaria, il tema dovrà essere affrontato e risolto,

non c'è dubbio che si pone un problema di opportunità politica. La mia tesi è che prima si affronta il problema, meglio è, ma si deve affrontare un problema sul lato dell'effetto di cassa facendo una valutazione su un punto estremamente controverso,

Presidente, molto spesso in quest'Aula il presidente Morando si alza per ricordare a tutti noi che si stanno esaminando argomenti complessi,

il relatore, senatore Legnini, ha più volte detto in Commissione che condivideva alcuni emendamenti dell'opposizione, ma che non poteva esprimere un parere favorevole perché era dubbia la copertura. Ciò vuol dire che se è dubbia la copertura non si può approvare un emendamento.

l'indebitamento è di competenza. Ora, da questo allegato conoscitivo, che ci è stato consegnato in fotocopia, ma che la Ragioneria generaledello Stato ha consegnato

Presidente, lei non può delegare al presidente Morando ciò che non è delegabile dal Presidente del Senato.

Non è possibile continuare così. Lei si deve assumere la responsabilità di dire se si può continuare di fronte a questa relazione tecnica che tale non è e non ci si può sentir dire né dal Presidente della Commissione

Presidente, vorrei innanzitutto che si comprendesse che l'emendamento 2.46, a firmato dal senatore D'Onofrio ed altri, non ha ad oggetto, come è stato detto - mi consenta il senatore D'Onofrio - un po' enfaticamente, problemi di grandissimo rilievo per la famiglia italiana. In realtà, si tratta di un problema molto contenuto,

Il senatore D'Onofrio, con l'emendamento, dice che sono cumulabili, a certe condizioni, tra coniugi e così via. È vero che durante l'espressione del parere ho detto quanto riportato dal resoconto, ci mancherebbe! Io, però, ho detto che, a mio modo di vedere, se il senatore D'Onofrio intendeva presentare un ordine del giorno, lo avremmo valutato. Presenti l'ordine del giorno e lo valuteremo! Personalmente, ritengo che nulla osti all'accoglimento di un ordine del giorno che preveda, nella prospettiva, la cumulabilità di queste detrazioni. Non mi ero espresso nel senso di un parere certamente favorevole ad un ordine del giorno che andrebbe, peraltro, letto ed esaminato. Quindi, ritengo che non sia conculcato alcun diritto, ma che vi sia che vi sia la possibilità di presentare l'ordine del giorno, di esaminarlo ed eventualmente accoglierlo. In ogni caso, se mi sono mal espresso, chiedo scusa al senatore D'Onofrio, ma la questione è tranquillamente risolvibile. Azzollini, non può intervenire su questo punto. Io ho comunicato, su richiesta di assunzione di responsabilità del Presidente, una decisione della Presidenza. Quindi, la Commissione è autorizzata a riunirsi e a riferire domattina su come questo argomento, toccato abbondantemente, possa essere affrontato.

Voglio ricordare che vi sono un problema ed un precedente specifici che la riguardano direttamente e che non hanno a che fare con la Commissione. Ciò che è insorto in Aula, signor Presidente, è un problema squisitamente politico. Quando, per la prima volta, ho posto in Commissione il problema di quell'emendamento, sollevando la mancanza di relazione tecnica, si poteva fare quel che lei ha detto: andiamo avanti, poi vediamo, il Governo provvederà. Oggi il problema è diverso perché non c'è la mancanza della relazione tecnica, ma c'è un documento, questa volta "bollinato" dalla Ragioneria, che evidenzia lo scoperto

Voglio dirle, signor Presidente, che a fronte della scopertura c'è un precedente preciso, che il senatore Morando non ha ricordato. Il Presidente della Repubblica

la Conferenza dei Capigruppo ha affrontato la questione emersa negli interventi svolti prima della sospensione

riprenderemo i nostri lavori con un intervento del Presidente della Commissione per vedere se su questo punto è stato fatto qualche ulteriore passo avanti, anche nei rapporti con le autorità istituzionali interessate. **Ripresa

abbiamo visto come sul caro mutui il Governo abbia a cuore la posizione di centinaia di migliaia di mutuatari o di famiglie, però nei vari interventi, sia del Governo, che dei relatori, non ho mai sentito pronunziare il termine

si è parlato di come procedere ad una elemosina per tutti coloro i quali pagano gli interessi, consistenti in una detrazione del 10 per cento dalla propria dichiarazione dei redditi, ripeto, non si è parlato di *spread*. Che cos'è lo *spread*? È la differenza che passa tra gli interessi pagati e la somma effettiva che centinaia di migliaia di mutuatari sono costretti a pagare alle banche per il rimborso spese delle banche e per l'utile della banca stessa. Cosa significa, signor Presidente? Che in aggiunta agli interessi pagati i mutuatari pagano

Basterebbe, signor Presidente, che il Governo proponesse una riduzione o una regolamentazione normativa dello *spread* per ridurre del 30 o 40 per cento l'importo della rata di mutuo. Credo che sia fondamentale ridurre la rata di mutuo o far applicare lo *spread* - se esso è dovuto comunque - in ragione percentuale degli interessi pagati stabilendo un tetto allo *spread* stesso. rappresenterebbe una riduzione sostanziale e rilevante rispetto agli interessi pagati e potrebbe essere perlomeno del 30 o 40 per cento della rata di mutuo che si paga. Questo credo che il Governo non lo ignori, ma non lo fa forse per proteggere determinati poteri che lo sostengono determinate espressioni bancarie alle quali non si vuole imporre per legge questa norma che certamente produrrebbe un vantaggio per tutti. Non rappresenta soltanto centesimi, ma talvolta il 100 per cento degli interessi pagati. Allora, questa è la nostra proposta: se veramente il Governo tiene a cuore

modo veramente si darebbe a tutti l'evidente dimostrazione che si vuole fare qualcosa per ridurre il caro mutui. Quindi, facciamolo e così veramente ci riteniamo oggi responsabili

ringrazio il relatore che mi ha chiesto di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, ma, dopo tanti anni di esperienza parlamentare, penso che gli ordini del giorno siano come il titolo di cavaliere nella Milano spagnola di Manzoni: non si negano a nessuno.

gente che si alza la mattina e va a lavorare all'estero. Si tratta di favorire i pensionati del lavoro frontaliero perché vedano una riduzione sulla loro tassazione. Chiedo all'Aula di esprimersi in maniera favorevole. È un problema annoso che va avanti dal 1999

nel merito, che sono intervenute infinite decisioni delle commissioni tributarie, che hanno riconosciuto la ruralità dei fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti dei soci conferenti. Inoltre, la legge di orientamento votata nella passata legislatura riconosceva la natura rurale dei fabbricati delle cooperative agricole. Quindi, ritengo che il relatore sia stato molto superficiale nell'esprimere

per quello che serve rivolgere appelli all'Aula, ho però visto qualche collega della sinistra prestare attenzione mentre illustravo questo emendamento. Esso tratta del modo sbagliato con il quale il nostro sistema tassa il TFR.

ricorrere a tutte le fonti di finanziamento possibili, ma andare a speculare su plusvalenze di enti *no profit* che sostanzialmente destinano ancora

Abbiamo cercato in tutti i modi di fare della famiglia un perno politico della finanza del Paese. Prendo atto che siamo stati sconfitti. Non credo che la maggioranza abbia vinto contro la famiglia. Se si illude di farlo, l'illusione dura poco. Le mie parole, da questo punto di vista, significano questo. Non mi rivolgo ai cosiddetti *teodem*. Non so cosa farmene. Mi rivolgo al partito egemone, al Partito democratico che sta nascendo: che sta nascendo: non si illuda che non capiamo che sulla famiglia la battaglia continua. Non è questione di singoli voti. È una finanziaria contro la famiglia e non è un caso. È contro la famiglia tutta l'impostazione politica di questa maggioranza. Mi chiedo fino a che punto questo Paese potrà tollerare questa continua volontà di scontro con un istituto fondamentale della nostra convivenza civile. Coloro che, all'interno del centro-sinistra si erano illusi di far valere alcuni di questi princìpi, princìpi, lo saranno per poco. L'illusione di queste persone non è quella rispetto alla quale le interviste potranno significare alcunché. Da questo momento in poi mi riprometto di non leggere più nessuna dichiarazione di questi cosiddetti *teodem*, sapendo che loro non contano nulla. Mi rivolgerò soltanto al Partito democratico nella speranza che possa trovare accoglienza questa nostra richiesta. *(Applausi

Presidente, vorrei ricordare che la sinistra ha votato contro i lavoratori frontalieri, contro i pensionati, ma

Esso chiedeva la deducibilità delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza. Siete, cioè, anche contro i portatori di *handicap*. Inoltre, siete contro la deducibilità delle spese sostenute per le rette degli asili-nido. Siete contro la deducibilità delle spese sostenute per le scuole materne, pubbliche o private; per quelle famiglie cioè monoreddito che, per far frequentare al figlio una scuola privata o pubblica, devono pagare rette fino a 300 euro al mese. Voi siete contro la deducibilità delle spese, per l'acquisto dei libri di testo, per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo. Non era mai avvenuto in questo Paese che la sinistra - il Partito democratico lo giudichiamo una sorta di *longa manus* del potere bancario, sul quale quindi non ci soffermiamo - votasse contro - votasse contro la deducibilità di queste spese è un'autentica vergogna, anche perché lo stesso centro-sinistra centro più che sinistra - fa uno sconto alle banche sull'IRES di molti punti. Allora fate pagare meno tasse alle banche usuraie che perseguitano i lavoratori a reddito fisso, che hanno comprato una casa, e siete anche contro la famiglia italiana e persino contro i portatori di *handicap*.

risorse, sia chiaro, su cui vogliamo discutere, ma che sono la condizione per garantire la possibilità che non entri in vigore la riforma Maroni a fine anno e per tutelare (anche se noi vogliamo ancora di più) i lavoratori italiani, siamo al paradosso. Noi votiamo dentro una maggioranza di Governo

non credo che la rivendicazione dell'orgoglio di appartenenza del collega Bobba gli faccia particolarmente onore. Noi voteremo contro questo articolo, perché questo articolo, perché pensiamo, nel nostro piccolo e con le risorse che avevamo a disposizione, di aver fatto qualcosa per la famiglia.

Viste le risorse per la cooperazione internazionale, che sono assai scarse, mi meraviglierebbe un non voto della maggioranza. Se ne è parlato tante volte della Tobin *tax* però la si rimanda sempre. Chiedo che questa volta essa venga introdotta e per questa ragione chiedo che tale

Buonasera, signor Presidente.

querele che possono scambiarsi i senatori come singoli cittadini, invito ad usare un linguaggio parlamentare. Nel rapporto fra colleghi, secondo me, questa è una regola che vale per tutti e che non prevede distinzioni, ovviamente.

rabbia per quello che ha denunciato il collega Castelli, il quale credo abbia ragione. Siete più agitati di quando fate le riunioni di maggioranza. Questa è l'Aula del Senato. Fateci parlare tranquillamente. Ha ragione chi sostiene il diritto della presidente Finocchiaro a parlare senza sentirsi rivolgere parolacce.

la restituzione del *fiscal drag* è una promessa incerta: io, invece, l'ho tradotta in una precisa proposta emendativa. Infatti, i lavoratori dipendenti perdono ogni mese da 50 a 100 euro a causa dell'anomala lievitazione del prelievo fiscale, versando più di quanto previsto dalla legge. In assenza del recupero del drenaggio fiscale richiesto da tutti i sindacati, si opera così un furto nelle tasche degli unici soggetti che pagano integralmente il fisco, con trattenuta alla fonte. Questo sì che sarebbe

alla sinistra più a sinistra del Partito Democratico) si opponga ad un emendamento che è parte della filosofia politica ed economica che esprime da sempre, cioè il recupero del drenaggio fiscale, che naturalmente penalizza in particolar modo i redditi dei

tutta quella sinistra: questa è la vergogna di chi voterà contro questo emendamento.

La copertura potrebbe essere rinvenuta in una norma che più volte è stata utilizzata ed accettata da parte della Presidenza, quella relativa alla conseguente riduzione proporzionale di tutti i capitoli di spesa, ad eccezione di alcuni che sono stati tipicamente sempre esentati da questo tipo di copertura, per così dire, In questo modo verrebbe meno l'obiezione (almeno per parte mia, ma penso anche nostra, del Gruppo di Forza Italia) sulla condivisione dell'obiettivo di eliminare il drenaggio fiscale, che non può che trovarci d'accordo.

La proposta è molto semplice; è una misura più volte preventivata anche nell'iniziativa della maggioranza, ma che non è mai arrivata Si tratta della tassazione delle rendite finanziarie al 20 per cento e della riduzione delle imposte sui conti correnti sempre al 20 per cento. Era nel programma dell'Unione, peraltro, ed anche nel testo iniziale della passata finanziaria, ma continua a perdersi per strada. L'emendamento 2.0.14 che la ripropone salvaguarda i piccoli risparmiatori con BOT sotto i 10.000 euro o con redditi sotto i 30.000 euro annui, che mantengono la tassazione al 12, 5 per cento. È inaccettabile che i lavoratori paghino il 33 per cento e gli speculatori il 12,5

delegata da collegare alla finanziaria. Chiedo al Governo di confermare questa disponibilità e questo impegno

Signor Presidente, mi associo alla richiesta del senatore Bonadonna, perché il Governo ribadisca in Aula l'impegno ad avere uno strumento normativo specifico su questo argomento,

debba tassare le rendite finanziarie in maniera armonica rispetto agli altri Paesi europei. Segnalo, infine, che i contenuti di questi emendamenti abbassano la tassazione dei depositi dal 27 al 20 per cento, dando un vantaggio per le famiglie, mentre per quanto riguarda i titoli e i loro rendimenti il 97 per cento sono in mano ai grandi intermediari finanziari.

è opportuna una conferma da parte del Governo, perché può essere utile nella sede dell'Aula, ma vorrei ricordare che in Commissione è stato approvato - e adesso sentiremo il Governo ribadire questo impegno un ordine del giorno per l'intervento sull'armonizzazione delle rendite finanziarie. Questo è un tema sul quale vi è stata, questa estate, una spregiudicata campagna di deformazione della verità. L'armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie, che era prevista anche nella risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria e che è sostenuta da autorevoli personalità e studiosi dei più diversi orientamenti, è una questione di civiltà vorrei dire al collega che non dovrebbe appartenere soltanto alla cosiddetta sinistra antagonista. Mi limito a segnalare che con il sistema attuale, senza bisogno di fare riferimento al rapporto tra redditoda lavoro e reddito da speculazione finanziaria, una persona ricca - per usare un'espressione semplice - se decide di utilizzare il suo capitale per investire e creare sviluppo, occupazione e benessere paga il doppio delle tasse che se lo gioca in Borsa o se si fa dare gli *stock option*. Abbiamo visto che è stato impossibile in questa sede far approvare questo testo, ma insisteremo, insieme al Governo, perché questa misura di civiltà fiscale sia approvata anche in Italia come in gran parte dei Paesi civili.

quando ero uno studente di legge, il professor Cosciani, grande maestro di scienza delle finanze, ci ha spiegato che quella delle rendite finanziarie è, per eccellenza, una tassazione che si trasferisce: non la paga il percettore della rendita, la paga chi paga l'interesse. Se tassiamo le rendite finanziarie, i tassi di interesse saliranno, perché i risparmiatori chiederanno di avere lo stesso tasso di interesse reale il paragone tra i tassi di interesse si effettua paragonando i tassi di interesse reale - e quindi bisognerà pagare un interesse più elevato. Conviene a noi, in questo momento di tensione del sistema produttivo, lavorare per l'innalzamento dei tassi di interesse? Per l'innalzamento dei tassi d'interesse sui titoli di Stato? Conviene a noi, in questo momento in cui il sistema bancario vacilla sotto l'impatto della crisi dei mutui *subprime* negli Stati Uniti, che ha innescato a catena altre vicende pericolose per la stabilità del sistema, indurre un ulteriore elemento di difficoltà e di crisi di sistema? Mi permetto di osservare ulteriormente: è questo il segnale che noi lanciamo ai contribuenti italiani, i quali non vogliono sentir parlare di tasse, neanche ove esse fossero eventualmente ragionevolmente proponibili perché il carico fiscale in Italia ha raggiunto ormai limiti intollerabili? È questo il messaggio che lanciamo ai contribuenti? È questo il messaggio che lanciamo ai risparmiatori? È questo il senso dello Stato, è questa la consapevolezza della complessità dell'economia italiana, è questo il livello di serietà, di correttezza e di onestà verso la pubblica opinione che manifestano questa maggioranza e questo Governo?

dà al Governo una indicazione su come muoversi, tant'è vero che il Governo ha accolto l'ordine del giorno della Commissione e ne confermo brevemente i contenuti. Anzitutto, l'idea è quella di arrivare ad un sistema di tassazione che faccia ordine nel rapporto fra orientamento di rendita o speculativo e capitale investito,

chiediamoci perché tanti capitali anziché essere investiti in modo produttivo prendano altre strade. La stessa cosa vale dal punto di vista del rapporto sulla tassazione dei redditi: le aliquote IRPEF arrivano fino al 43 per cento e il 12,5 è chiaramente troppo conveniente. Se non ricordo male, il quotidiano «Il Giornale» ha svolto recentemente un'inchiesta in cui ha sottolineato che i redditi di una ventina di persone, nell'arco di dieci anni, hanno portato più o meno a 5 miliardi di introito. Non è poco per un numero così ristretto di persone. Mi pare del tutto evidente che la tassazione di quegli introiti da *stock option* e

è un provvedimento che il Governo inglese ha preso nei giorni scorsi; è un orientamento che riguarda anche altri Paesi, tant'è vero che l'aliquota sulle rendite finanziarie in Europa sta mediamente cento. Non è vero che questo porterebbe a chissà quale risultato dal punto di vista dei rapporti nella tassazione sulle rendite perché saremmo esattamente in una media di natura europea. Il di più - ci potrebbe essere un di più tra la diminuzione dei conti correnti (oggi al 27 per cento) e l'elevazione dal 12,5 magari al 20 delle rendite finanziarie - potrebbe tranquillamente essere riutilizzato o, meglio, dovrebbe essere riutilizzato a fini di riduzione della tassazione di chi oggi paga troppo anche perché c'è un settore della società o dei redditi che pagano troppo poco.

sede. Non dimentichiamo, infatti, che questo è un argomento di qualche complessità e merita di ritornare nell'ambito del disegno di legge delega, che è all'esame della Camera, che affronta la tassazione dei fondi mobiliari italiani ed esteri - oggi quelli italiani sono sfavoriti - perché, in quell'ambito, si potrebbe trovare un'opportuna sistemazione di entrambi gli argomenti. tassazione dei fondi mobiliari italiani ed esteri nello stesso modo e, allo stesso tempo, alla tassazione ad un livello più accettabile ed accettato delle rendite finanziarie. Poiché l'argomento ha una certa complessità e deve essere affrontato con strumenti adeguati, l'ordine del giorno che il Governo ha accettato, e che confermo nella sua accettazione, indica al Governo di riprendere il cammino esattamente nel disegno di legge delega

perché essi rappresentano un modo organico di risolvere i problemi della famiglia che la nostra parte politica propone. Prima si è scatenata una polemica, ma posso assicurare che la memoria non è corta e che durante la passata legislatura sono state prese molte misure molto interessanti sulla questione. Ciò è del tutto innegabile e talvolta negare i fatti non è positivo. Noi continuiamo su questa strada e offriamo la possibilità al Governo di effettuare una politica sulla famiglia particolarmente incisiva. Voglio ricordare, in particolare per l'emendamento 2.0.23, che proponevamo la cessazione della partecipazione statale in Sviluppo Italia, che è una società che, come tutti sanno, fa molta Italia e poco sviluppo.

Lo stesso vale per le misure di sostentamento per i nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti, e anche a questo proposito contestiamo all'altra parte il

di questi emendamenti configura un'alternativa politico-programmatica per i nuclei familiari che ci pare assolutamente coerente. Per questo ne chiediamo l'approvazione e

è detto che il Senato invita il Governo a rivedere l'attuale normativa. Quindi, non c'è nulla da attenuare. Se il relatore ritiene che invitare il Governo a rivedere la normativa sia troppo duro, esprima parere contrario e io chiederò che l'Aula voti

"invita il Governo" e quindi l'iniziativa legislativa è nella potestà del Governo, così come sarà nella potestà del Parlamento decidere se l'iniziativa legislativa dovrà avere un'altra piega o no.

premesso: che con l'emendamento 2.46 si è chiesto il cumulo dei benefici a favore dei contratti di locazione per entrambi i coniugi, al fine di favorire la famiglia; che la proposta del Governo invece propone il godimento del beneficio per nuovi contratti di locazione in egual misura sia che si tratti di famiglia che per *single*, invita il Governo a rivedere l'attuale normativa a favore dei contratti di locazione rivolti a nuclei familiari.

Presidente, per la verità, avevo chiesto di intervenire sull'emendamento 2.0.31, pur credendo anch'io che sia inammissibile in quanto incostituzionale. Tuttavia, proporrei al presentatore di trasformarlo in un ordine del giorno,

poi ricostituiti dal Governatore a capo della Banca d'Italia dal 1993 al 2005 e che oggi la Banca d'Italia ha un *surplus* di riserve monetarie. Quindi, se il Parlamento approva un ordine del giorno e pone il problema alla Banca d'Italia, che in autonomia possa verificare se parte delle riserve in esubero possono essere utilizzate per ridurre il debito pubblico, personalmente sono d'accordo, tanto più che l'attuale Governatore, che non ha meriti storici nella ricostruzione di queste riserve, nel passaggio delle audizioni in finanziaria, ha mostrato una linea di rigore ed ha denunciato a più riprese che il debito pubblico e la spesa pubblica sono da controllare con molta attenzione.

Per limitare la facoltà dei Paesi di mettere ingenti masse d'oro sul mercato, il Consiglio d'Europa, su suggerimento della BCE, in convenzione con tutte le 14 banche europee Regno Unito, che, come è noto, non usa l'euro), stabiliscono che vi è una convenzione, sino al 2010, per cui si possono mettere sul mercato al massimo 500 tonnellate di oro l'anno e queste somme vanno a riduzione del debito dei Paesi. Non capisco che cosa si viola nella Costituzione o quale norma europea, a meno che non l'abbiano violata lo stesso Consiglio d'Europa o la BCE che,